Nel corso della seduta di ieri la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea. Poiché l'estensore del parere, senatore Mancuso, non intende intervenire,

disposizioni interessate dalle nostre censure di costituzionalità sono contenute esattamente negli articoli 20 e 21 del decreto-legge in conversione, che nella sostanza dispongono la modifica di taluni fondamentali aspetti della normativa vigente in materia di funzionamento del modello cooperativistico del credito fondato sulla cosiddetta democrazia economica, che è proprio il *modus operandi* delle banche di credito cooperativo, delle banche popolari e delle allora casse di risparmio. Si tratta di un modello radicalmente diverso da quello tipico degli istituti di credito organizzati nella forma societaria delle società per azioni, il cui principio fondante (un'azione, un voto) è opposto alla democrazia economica tipica del credito cooperativo, che si fonda sul principio del

a struttura cooperativa in difficoltà - ovviamente lo prevedono in termini generali e non certo per il caso MPS - ne modificano (e qui viene la norma che noi censuriamo) gli aspetti essenziali, ad esempio tramite la sostituzione del voto capitario con quello per azione, o anche modificando l'accesso alla compagine sociale in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2527 e 2528 del codice civile. Tali interventi, pur essendo rivolti a tutelare l'eventuale investimento statale - come evidenziato nella relazione introduttiva, in cui si sostiene che gli istituti della cosiddetta democrazia economica non sono idonei a garantire quell'investimento - sono, a nostro avviso, palesemente incostituzionali. È noto a questa Assemblea, infatti, che lo strumento della decretazione d'urgenza debba contenere misure di immediata applicazione, così come statuito dal comma 3 dell'articolo 15 della - più volte citata - legge n. 400 del 1988, pacificamente considerata di rango costituzionale. È evidente che tali interventi siano tutt'altro che di immediata applicazione, sostanziando invece una riforma organica del credito cooperativo, con il pretesto dell'ipotetico intervento statale. Questo tema è all'esame del Parlamento e anche del dibattito politico da mesi e mesi: il Governo cerca di introdurre in pillole questo tipo di riforma del credito cooperativo, strada percorsa dal Governo Renzi con la riforma delle banche popolari recentemente già censurata dalla Corte costituzionale. È ormai consolidata la giurisprudenza della Corte, secondo la quale un decreto-legge che contenga norme, quali quelle di cui agli articoli 20 e 21, non immediatamente applicabili, configura un vizio di eccesso di potere del legislatore governativo;

circa il corretto uso del decreto-legge come fonte del diritto e strumento di governo, affinché il ricorso ad esso non trasmodi in eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica di tale strumento, di cui all'articolo 77 della Costituzione. Per cogliere la pregnanza della giurisprudenza della Corte in materia di decretazione d'urgenza, che con questa pronuncia si consolida ulteriormente in termini univoci nella direzione di evidenziare i limiti formali e sostanziali a tale potere, non è irrilevante come la stessa Corte abbia evidenziato il fatto che il decreto-legge si collochi come fonte del diritto in quanto frutto primario di una scelta dell'Esecutivo e non del Parlamento. Per tale ragione la Costituzione ne ha circoscritto l'adottabilità tanto alle circostanze di fatto di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, quanto nell'ambito dei limiti formali che qualificano la forma di governo in vigore, che si imperniano sul rilievo del procedimento legislativo ordinario presso le Camere, quale sede ordinaria per la posizione del diritto primario, soprattutto quando esso rechi discipline di tipo ordinamentale.

segnalare l'incostituzionalità anche solo di alcune parti di un decreto-legge in conversione. In questo senso va il nostro intervento a sostegno dei rilievi di incostituzionalità mossi al decreto.

Signor Presidente, anche noi sosteniamo i presupposti di incostituzionalità di questo decreto-legge e muoviamo queste osservazioni basandoci su un'argomentazione molto semplice. Il Governo negli ultimi tempi ha varato tutta una serie di provvedimenti provvedimenti (definiti decreti salva banche, salva risparmio eccetera) con trattamenti evidentemente diversi rispetto ad azionisti e obbligazionisti delle banche coinvolte. Ci sono stati dei primi provvedimenti nel novembre del 2015 che tendevano a salvare - così è stato detto - quattro banche in grave dissesto.

equità di trattamento nei confronti di risparmiatori di banche coinvolte in dissesti finanziari e che inoltre si renda necessario l'accertamento delle responsabilità (e su questo si dovrà muovere la Commissione d'inchiesta, che speriamo venga finalmente varata); costituzionalmente sostenibile che ci siano azionisti o obbligazionisti di alcune banche che hanno perso tutti i loro risparmi, altri che vengono parzialmente indennizzati, altri che vengono tutelati con formule nuove e innovative come quelle contenute nel decreto-legge con il quale si chiede nuovamente un intervento d'urgenza

Oggi nel nostro Paese tutti i cittadini italiani hanno la certezza che i propri risparmi, i risparmi di una vita, non sono al sicuro rispetto ad errori o addirittura a

a tutela di altri istituti creditizi, con provvedimenti nuovi e improvvisati, che non avranno niente di equo e soprattutto di uniforme rispetto ai provvedimenti precedenti. Chiediamo uniformità di trattamento e una tutela per risparmiatori, azionisti e obbligazionisti che sia omogenea in ogni caso. Non ci possono essere trattamenti di serie A o di serie B; la Costituzione non lo permette e per questo chiediamo chiediamo naturalmente un voto del Parlamento che prenda atto di questa situazione ormai fuori controllo per responsabilità precise del Governo precedente e di quello attuale (che ne è una fotocopia), e che non sa più dove andare a parare.

abbandonati a sé stessi, in balia degli eventi, senza alcuna certezza e con un'unica grande preoccupazione, cioè che i risparmi di una vita possano essere cancellati nel giro di una notte con un decreto-legge che non salva certamente i loro risparmi, ma che può salvare gli istituti bancari che cerca di coprire le responsabilità di chi ha determinato queste situazioni in un crescendo ormai intollerabile. Mi auguro che il Parlamento prenda atto di questa situazione ormai fuori controllo e voti una incostituzionalità che è evidente, palese, certa e deve essere semplicemente ratificata con il voto del Parlamento. *(Applausi dei

una sforbiciata al risparmio della banca da parte della BCE per ben 13 miliardi di euro), il Governo Renzi ha voltato la testa dall'altra parte, preferendo continuare la battaglia

ci troviamo di fronte ad una risposta a questo punto assolutamente tardiva. Non solo, ma all'interno di questo decreto-legge vi è una serie di provvedimenti

Oltretutto, la risposta del Governo sembra ancora una volta sempre più incentrata sul salvataggio delle banche (e magari, nel caso specifico, del MPS), senza porre al centro la vera questione che è

manca assolutamente un seppur minimo accenno alle responsabilità che ci hanno portato alla situazione attuale; responsabilità da cui non risultano certamente esenti esponenti del precedente e dell'attuale Governo, che non hanno saputo agire con la necessaria tempestività al fine di tutelare il risparmio. Ieri abbiamo assunto la decisione di estendere l'urgenza a tutti i

sulla trasparenza, perché tutti gli italiani hanno il diritto di conoscere i nomi di tutti i maggiori debitori insolventi. Questo ha molto a che fare anche con i presupposti di costituzionalità, perché è evidente a tutti che rischiamo di trovarci di fronte a trattamenti diversi e quindi ad una tutela non adeguata soprattutto dei piccoli risparmiatori.

il cosiddetto *bail in*; nel contempo, il Governo Renzi emette un decreto-legge per la risoluzione di quattro banche.

avrebbero portato comunque a un peggioramento della fiducia dei cittadini italiani nel nostro sistema bancario.

il sistema bancario italiano, ossia quel tessuto che dovrebbe far crescere l'economia e i cittadini stessi, potrebbero avere qualche dubbio sull'investirci. avevamo pertanto chiesto di mettere subito in chiaro quali erano le procedure che si potevano effettuare attraverso la direttiva BRRD per intervenire pubblicamente. C'è stato risposto che non era possibile.

Quest'Assemblea diceva che non si trattava di piccoli risparmiatori, ma di investitori. Però, a un certo punto, la maggioranza si è resa conto che forse avevamo ragione noi e che i piccoli risparmiatori sono stati truffati.

a luglio 2016, escono i risultati degli *stress test*. Noi sapevamo già in anticipo che il Monte dei Paschi di Siena non avrebbe retto agli *stress test*, perché il percorso degli ultimi anni della banca aveva comunque evidenziato una mancanza di patrimonio e di liquidità; infatti, il titolo stava crollando. Al Governo però non interessava rimettere in piedi il sistema bancario: gli serviva solo un'arma di ricatto. Infatti, nella

Si arriva al *referendum* e si perde, ma la questione della Monte dei Paschi era già nota; non c'era però la necessità e urgenza in quel momento perché tanto si aspettava.

questo Governo pensa alla necessità e all'urgenza del Paese, oppure alla propria necessità e urgenza di rimanere al suo posto per continuare a coprire quelle amministrazioni bancarie e quella

di farvi riprendere il contatto con il territorio. Forse non siamo stati abbastanza incisivi o forse voi siete troppo sordi, ma questo decreto-legge non è necessario e urgente.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, senza nulla togliere all'autorevolissima presenza di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari, mi sarei aspettato oggi la presenza del ministro Pier

che sono apparsi come un florilegio delle sue dichiarazioni del tutto rassicuranti sulla situazione del Monte dei Paschi. Per tacere di quanto l'ex presidente del Consiglio Renzi ha detto più volte, in particolare un anno fa, il 22 gennaio 2016: 22 gennaio 2016: il Monte dei Paschi è risanato, ora investire è un affare. Forse avrebbe dovuto far seguire queste dichiarazioni dalla consueta formuletta: "la presente non costituisce sollecitazione al risparmio o all'investimento su questi titoli". un bancario che facesse un'affermazione di questo genere, senza precisare quanto ho sopra specificato, rischierebbe sanzioni penali. Invece abbiamo un ex Presidente del Consiglio che ha detto di investire in questa banca e chi ha investito si è ritrovato il capitale ridotto più o meno del 90 Pertanto, quanto dico non è solo strumentale a parlare di fatti passati, le cui conseguenze, in realtà, sono pienamente presenti in questo decreto, ma sottolinea il primo difetto di questo decreto e cioè che giunge tardivo.

anziché 20 miliardi di euro sarebbe stata necessaria una somma molto inferiore. Un articolo di Marcello Esposito su «la Repubblica», non proprio un giornale antigovernativo, ricordava qualche giorno fa che, negli ultimi sei mesi, il Monte dei Paschi ha perso 14 miliardi di depositi,

Inoltre, l'accoglimento eccessivamente affrettato e non sufficientemente spiegato del famoso meccanismo del *bail in* ha fatto sì che molti, specialmente dalle banche che avevano il sentore di qualche difficoltà, siano fuggiti. Il risultato è che le banche che già erano in difficoltà sono finite in grave difficoltà e ora tocca al contribuente ripararle: davvero un errore gravissimo che dimostra l'insufficienza fondamentale della politica bancaria del Governo precedente e, per quanto di competenza, del Governo presente. Ecco perché avrebbe dovuto essere presente il Ministro dell'economia, che invece forse sta facendo qualche altra dichiarazione

ha contribuito a far sì che oggi possiamo parlare di un decreto. Modificarlo in meglio o in peggio sarà poi compito, in parte, del Governo che, purtroppo, non ha ritenuto di consultare coloro che si sono coinvolti in questa presa di responsabilità e, in parte, del lavoro che faremo in queste settimane. Ricordo, però, che trattandosi di decreto-legge, nel frattempo esso è in vigore. Pertanto, se ci sono degli errori, essi si riflettono fin da ora nella realtà e sarà difficile correggerli. Un altro problema di questo decreto è la disparità la disparità di trattamento con le altre banche che si sono trovate in difficoltà; una disparità molto grave, denunciata, per esempio, dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il quale ha

In secondo luogo, la situazione può dare luogo a dei ricorsi per evidente vizio di costituzionalità a fronte dell'articolo 3 della Costituzione, che prevede l'eguaglianza tra i cittadini

radicale della Costituzione per risparmiare 50 milioni, e poi qui si parla di 20 miliardi come se fossero noccioline; 20 miliardi che rischiano di aumentare con questa disparità di trattamento. questo è un difetto davvero notevole del provvedimento in oggetto, che bisognerà sicuramente prendere in esame. Altro problema fondamentale di questo decreto-legge è che in esso non vi è traccia di misure che impongano al Governo di rendere conto di come questa somma verrà impiegata. Si parla di 20 miliardi di euro che escono subito dal bilancio dello Stato, con una formula curiosa. Mentre, ordinariamente, quando c'è un fondo di garanzia l'uscita per il bilancio dello Stato avviene quando questa garanzia deve davvero intervenire. Qui, invece, i 20 miliardi escono subito, e quindi aumenta il debito pubblico con tutte le conseguenze anche sulla strategia finanziaria del nostro debito, e poi il Governo li utilizzerà. Noi sappiamo che la cifra relativa al Monte dei Paschi sarà compresa fra i sei (speriamo) e gli otto (temiamo) miliardi, ma gli altri?

peraltro vengono in gran parte lasciate alla discrezionalità di scelte che dipendono dal Governo o vengono compiute direttamente dal Governo. La situazione di emergenza impone almeno in parte queste scelte, ma è fondamentale che il Governo ne riferisca e ne spieghi i criteri. altro aspetto che vogliamo sottolineare è che è necessario introdurre (e riteniamo questa la sede più opportuna) norme che impongano di rivelare i nomi e le identità di società o di privati che siano grossi siano grossi debitori insolventi delle banche, che poi vengono aiutate a spese del cittadino. I dipendenti dello Stato, gli eletti dal popolo devono rendere conto dettagliatamente di quanto prendono. Lì parliamo di decine di migliaia di euro. Poiché qui parliamo di miliardi, sarà bene essere almeno altrettanto rigorosi. Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare che se ci sono stati dei prestiti dei prestiti la cui restituzione è in sofferenza, vi è anche qualcuno che questi prestiti li ha concessi e che è più colpevole, perché ancora più responsabile. Di questo sarebbe bene avere contezza. Non è possibile, ad esempio, che in questo decreto si stabilisca che si diano per truffati tutti coloro che hanno comprato delle obbligazioni subordinate - e questo è anche opinabile - senza che però ci sia il truffatore. Se lo Stato deve intervenire a rifondere coloro che hanno comprato dei titoli che, seguendo il codice civile, oggi hanno perso moltissimo del loro valore,

ieri si era espresso a favore della proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, che ovviamente è l'oggetto della conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Troppe vicende che hanno riguardato quell'istituto sono ancora avvolte nel mistero, compreso l'apparente suicidio (ma poi è stato veramente così?) di un dirigente precipitato da Rocca Salimbeni.

ma la vicenda è molto più complessa. Riguarda legami che risalgono ad un tempo ancora più lontano e che hanno investito l'intero gruppo dirigente del Partito comunista, poi PDS, DS ed ora PD tanto a livello locale che nazionale. Alcune operazioni, infatti non potevano essere poste in essere se non vi fossero state complicità diffuse

Vincenzo Visco - intervenne pesantemente per indirizzare la nomina del nuovo presidente dell'istituto nella persona di Giuseppe Mussari: unico non senese ad assumere quella carica che nei 500 anni precedenti era spettata di diritto ad un cittadino del luogo.

sarebbe meglio dire sotto maglietto. Si illumineranno le manovre iniziate fin dagli anni Settanta ad opera di personaggi poco noti al grande pubblico, ma non alla nomenclatura di quel partito. Fu Silvano Andriani, uno dei consiglieri della banca, a far conoscere, a Roma, le potenzialità di un istituto che, negli anni precedenti, aveva avuto solo un'importanza locale. Silvano Andriani, prima di essere eletto come senatore, era stato il segretario del CESPE: chi ha i capelli bianchi come me ricorda che era il centro studi di politica economica del Partito comunista. Un vivaio di giovani quadri dove almeno due ministri attuali Pier Carlo Padoan e Claudio De Vincenti - compivano i primi passi. Questo per dimostrare quanto sia lunga la tela di quella storia. mi soffermo sulle vicende più recenti che questo decreto ben esplicita. Negli ambienti finanziari si parla, con insistenza, di un possibile scambio, a livello europeo. La Commissione che chiude un occhio sulle misure di salvataggio di salvataggio predisposto, in aperta violazione delle norme del *bail in* per evitare di accendere i fari sul vero grande malato d'Europa, vale a dire la Deutsche Bank con il suo carico di derivati, la cui valutazione è stata lasciata alla discrezionalità della stessa banca, mentre alcune operazioni sono state valutate in modo improprio per rafforzare la sua consistenza patrimoniale. Già questo accenno dimostra come il problema degli assetti del sistema bancario italiano vada ben oltre il caso del Monte dei Paschi di Siena. Ecco perché in questo momento

proceduto al rimborso dei debiti contratti e che di conseguenza hanno alimentato i *non performing loans*, che rappresentano la palla al piede dell'intero sistema bancario italiano. Diceva un mio collega di Gruppo, il senatore Milo, che bisognerebbe nazionalizzare le imprese che hanno preso i soldi dallo Stato e non li hanno restituiti, non dare i soldi al Monte dei Paschi per coprire questi buchi che hanno creato dolosamente. I problemi lievitano

si indicava con grande preoccupazione che le banche italiane avevano crediti in sofferenza per un valore che le collocava al terzo posto nella classifica internazionale, subito dopo la Grecia e l'Irlanda. Si tratta di una denuncia che evidentemente non ha scosso chi invece doveva preoccuparsi. Queste sono solo alcune ragioni per per dimostrare la necessità di estendere il presente decreto a tutto il sistema bancario, non solo al Monte dei Paschi. Troppe cose rimangono misteriose, a partire da una vigilanza, quella della Banca d'Italia, che ha operato con discrezionalità e intermittenza: feroce feroce con alcune piccole banche - ne cito una, il Credito cooperativo fiorentino - ma del tutto comprensiva e ovviamente complice in tutte le altre situazioni, compreso il Monte dei Paschi di Siena, al punto da determinare i risvolti di carattere giudiziario poi terminati Nella nostra proposta, quindi, oggi riteniamo che il nostro obiettivo coincida con quello indicato dal presidente dell'ABI: rendere noti i nomi dei grandi profittatori di una risorsa come il risparmio, specificatamente tutelato dall'articolo 47 della nostra Costituzione. Ecco perché il nostro voto sarà contrario, proprio perché il testo non rispetta quest'articolo 47. Dobbiamo separare le mele marce (poche) da quelle buone (tante) Siamo infatti convinti che la maggior parte delle banche italiane sia solida e in grado di svolgere la sua funzione essenziale, che è quella di finanziare lo sviluppo economico del Paese. preservare tale funzione, però, è necessario non solo mettere in fuorigioco chi si è approfittato della pubblica buona fede, ma far emergere prima che sia troppo tardi quei problemi ai quali si può ancora provvedere. Un compito, questo, che non può essere lasciato ad *Authority*

di votare favorevolmente ai presupposti di necessità e urgenza di questo provvedimento fossimo tutti, o quasi, d'accordo. Se non c'è stata totale condivisione, sicuramente non ci sono state le riflessioni e gli interventi che oggi ho ascoltato in Aula, che riguardano più che altro il merito del provvedimento. Poco ho sentito dal punto di vista delle motivazioni che possono essere ostative circa l'accoglimento dei presupposti di necessità e urgenza. urgenza. Ritengo che la discussione di oggi sia stata un po' anticipatoria del dibattito successivo, però noi ora ci dobbiamo limitare all'approvazione e all'accoglimento

serie. Al Capo I del provvedimento è disciplinata la procedura per la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di banche aventi sede legale in Italia. Il Capo II riguarda gli interventi di rafforzamento patrimoniale, e se questi interventi non si fanno con la dovuta ritengo che si possa anche vanificare l'intervento del Governo in aiuto e supporto al sistema bancario. ci sia la necessità di una riorganizzazione, di una revisione e di una riflessione totale sulla necessità - così come è stato detto ieri - di verificare il comportamento di chi ha le responsabilità di monitorare

dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012

Signor Presidente, l'Azerbaijan, che è membro del Partenariato Euro-Atlantico, occupa un'area di grande importanza strategica e politica, che costituisce però anche un crocevia di traffici illeciti, i cui proventi alimentano spesso attività criminali di vario tipo sul territorio europeo. Nell'ambito delle intese bilaterali con l'Azerbaijan, il Parlamento ha recentemente autorizzato un disegno di legge - ora in attesa di pubblicazione - relativo ad un Accordo di cooperazione nel settore della difesa.

individua e definisce le diverse tipologie di reati (dalla criminalità organizzata al terrorismo, fino al traffico di stupefacenti e di esseri umani) cui si applica. La cooperazione prevede lo scambio di informazioni e di esperienze, la ricerca di latitanti e di persone scomparse, l'identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione e l'applicazione di mezzi tecnologici moderni per il contrasto ai traffici di persone e di migranti. Le richieste di assistenza possono essere respinte solo se compromettono la sicurezza nazionale o risultano in contrasto con la legislazione nazionale. particolare, definisce i limiti e i livelli di protezione relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi nell'ambito della cooperazione bilaterale, disponendone un utilizzo per i soli fini dell'Accordo, salvo diverso consenso fra le Parti. Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 60.000 euro annui. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, ed è anzi in linea con le Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata. In conclusione, la Commissione mi autorizza a proporre all'Aula l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in

le spiegazioni necessarie all'Assemblea per comprendere la portata di questa ratifica. Mi limito a dire che abbiamo un orientamento favorevole per quanto riguarda la votazione finale e in sede di dichiarazione di voto fornirò le motivazioni.

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia e tra la Repubblica Italiana e lo Stato del Qatar; questo perché tutti e quattro i provvedimenti per

il testo in esame riguarda un aspetto importante, come richiamava il collega Amoruso, cioè la collaborazione dell'Italia nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare con riferimento alla prevenzione, alla scoperta ed alla repressione dei reati e all'individuazione dei criminali. Di qui, un'azione comune tra le autorità italiane e del Governo dello Stato del Qatar. Il testo si compone di un preambolo e di 11 articoli e mira a definire uno strumento giuridico che regolamenti la collaborazione di polizia bilaterale sotto il profilo strategico ed operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi. Nel definire gli obiettivi del *Memorandum*, l'articolo 1 menziona la collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalità, in generale e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati, nonché l'individuazione dei criminali, richiedano un'azione comune tra le autorità dei due Paesi. L'Accordo è finalizzato, in particolare, a contrastare, attraverso una cooperazione di polizia, i traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di armi, il terrorismo, la criminalità organizzata, l'immigrazione illegale e altri reati in qualche modo riguardanti il crimine organizzato. La cooperazione implica lo scambio delle informazioni e l'assistenza nello sviluppo scientifico e tecnico delle indagini. Gli articoli seguenti disciplinano i casi in cui le richieste di assistenza possano essere rifiutate, lo scambio di riunioni e visite e le misure di tutela per la protezione dei dati personali. Le autorità competenti sono il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e il Dipartimento per la cooperazione internazionale per il Qatar. disegno di legge consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri ed all'entrata in vigore del testo. Gli oneri complessivi sono di circa 50.000 euro annui. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità. Il testo tiene conto delle disposizioni contenute, fra le altre, nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

vede tutti schierati dalla stessa parte ma, poiché siamo in un momento delicato, bisogna prestare attenzione a provvedimenti come questo e soprattutto bisogna capire quali sono i soggetti con cui ci si interfaccia, quando vengono siglati accordi di questo tipo. Non si tratta di provvedimenti di serie B, ma di provvedimenti che hanno un impatto sui cittadini. Una ratifica di questo tipo ha sicuramente una portata positiva per quanto riguarda

in altre aree del mondo. È necessario capire se, effettivamente, chi firma con noi un accordo è scevro da questo tipo di sostegno a soggetti che hanno intenzioni ostili oppure vi è stata una una connivenza, che deve essere assolutamente condannata e non deve più esserci in futuro. Quando si parla di Qatar, si parla di uno Stato che sostiene la diffusione della religione islamica in tante altre parti del mondo, oltre ai Paesi dove essa si è originata e spesso lo fa mettendo a disposizione tantissimi soldi, tanti milioni di euro. Anche in proposito bisognerebbe capire quali siano le intenzioni reali: si tratta solamente di agevolare

evidenziando però che la portata del provvedimento è sicuramente positiva e che ci troviamo di fronte ad un Paese che ha dato dei segnali che, almeno nell'ultimo periodo, fanno ben

in modo molto più puntuale le perplessità poc'anzi espresse e ribadisco il voto di astensione del nostro Gruppo. Signor Presidente, l'illustrazione del collega Compagna è stata puntuale e dettagliata. Non c'è dubbio che l'argomento, anche alla luce delle riflessioni che ha sollevato il collega Stucchi, vada nella direzione di una maggiore conoscenza e di un maggior approfondimento. Tuttavia, proprio per dare migliori risposte in futuro credo sia opportuno non solo condividere, ma anche sostenere convintamente questo disegno di legge e, in particolare, quanto contenuto all'articolo 1.

i temi che si trattano tra i due Stati sono la collaborazione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il terrorismo, la criminalità organizzata, tutti e di contrabbando, il riciclaggio, i reati connessi alle carte di credito, i reati informatici e suInternet, i reati commessi nei porti, aeroporti e altri varchi e l'immigrazione clandestina.

per annunciare il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento. Le finalità, come ha detto il presidente Sangalli, sono buonissime, il problema è il soggetto con cui l'Accordo viene fatto. Credo che, per le implicazioni che ci sono state da parte di quello Stato con organizzazioni

L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a sviluppare una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, con particolare riferimento all'immigrazione illegale, alla tratta degli esseri umani e al traffico di sostanze stupefacenti. L'intento è di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sul piano strategico e operativo, nonché di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla pubblica sicurezza. L'Accordo, composto da un preambolo e da 17 articoli, individua nei rispettivi Ministeri dell'interno le autorità responsabili dell'attuazione dell'intesa. Dopo aver specificato gli ambiti di competenza per territorio, l'intesa definisce le modalità della cooperazione transfrontaliera prevedendo lo scambio di informazioni, i collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni, l'armonizzazione dell'attività operativa, istruzione e formazione professionale. I successivi articoli dell'Accordo disciplinano uno scambio di funzionari di polizia, gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e il coordinamento di attività operative. Un capitolo specifico è dedicato alla protezione della riservatezza dei dati personali. Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 120.000 euro annui, ascrivibili alle spese per la diaria e per il distacco di breve termine del personale coinvolto, nonché per l'attività di formazione e istruzione. Segnalo all'Assemblea che la Commissione affari esteri ha approvato due emendamenti al testo originario seguendo le indicazioni formulate dalla competente Commissione bilancio per spostare la copertura finanziaria al 2017 e per aggiornare le norme sulla copertura alla riforma delle legge di contabilità entrata in vigore lo scorso settembre. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e i relativi protocolli. In conclusione, signor Presidente, si propone l'approvazione del provvedimento in

Signor Presidente, voglio dire due parole in merito all'Accordo in esame, partendo dalla crisi siriana, che può essere definita, senza ombra di dubbio, la madre di tutte le emergenze migratorie in Europa dal 2011 in poi, oltre alla crisi libica, che sarebbe meglio definire l'aggressione militare a un Paese sovrano con l'obiettivo di annientare le istituzioni e favorire il caos. crisi influiscono sui flussi migratori, ma in questo caso mi riferirò alla crisi siriana per ovvie ragioni di geografia dei flussi migratori verso l'Europa. Questa crisi ha generato un enorme flusso di profughi, dei quali un numero sempre maggiore si dirige in Europa. Di fronte alle problematiche generate da quanto appena illustrato, la posizione politica della Croazia e degli altri Paesi dell'Est Europa è stata di totale contrasto alla ripartizione delle quote migranti, facendo di fatto pesare l'accoglienza su Paesi come il nostro e la Grecia. La Croazia, inoltre, ha più volte chiuso le proprie frontiere, creando di fatto situazioni di emergenza significative sia per gli Stati limitrofi, che per l'Europa in generale. problema, signor Presidente, non è dunque l'accordo in sé, ma il segnale politico che diamo alla Croazia, in un momento in cui questo Paese, in contrasto con altri, attua frequenti chiusure delle sue frontiere e a livello europeo gioca in un campo avverso al nostro

ed è stato più volte terreno di corruzione e malaffare, come ben sappiamo e come molti colleghi del PD ben sanno, con i casi di mafia capitale e del CARA di Mineo. di Mineo. Signor Presidente, parliamo tanto di immigrazione irregolare dal Mediterraneo (circa 150.000 arrivi in media all'anno) quando dalle Repubbliche dell'Est Europa ogni anno milioni di persone si spostano da aree dove il salario di un operaio è di circa 200 euro: mi pare chiaro che qualcosa non funzioni. Voi la chiamate integrazione, ma a mio avviso siamo di fronte ad un processo migratorio ben più imponente che sta abbattendo, una dopo l'altra, tutte le conquiste sociali e lavorative faticosamente raggiunte con la lotta dei nostri nonni e dei nostri padri. padri. Le reiterate azioni di chiusura della frontiera da parte della Croazia e il sostegno ad una proposta politica europea di gestione delle quote di redistribuzione dei migranti che danneggia in maniera sia diretta che indiretta l'interesse italiano sono le ragioni che portano il Movimento 5 Stelle a votare contro questo Accordo e invito i colleghi degli altri Gruppi politici a unirsi e dare un segnale politico inequivocabile

uno dei primi passi di una politica molto attenta rispetto a tutta l'area dei Balcani, sia per quanto riguarda i flussi di migrazione, sia in vista di un processo di stabilizzazione dei Balcani stessi.

*relatore*. Signor Presidente, il collega, senatore Amoruso, ha già delineato il senso e le finalità di questo provvedimento, ma in vista di una valutazione più dettagliata dirò che l'intesa in esame risponde all'esigenza di migliorare la cooperazione operativa tra le forze di sicurezza dei due Paesi,

sono inclusi la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, la migrazione illegale, la tratta di persone e quella di armi, nonché i reati di natura economica e il terrorismo. Il testo definisce quindi le modalità per lo svolgimento della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, lo scambio di informazioni e di prassi operative, lo svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative informative ed investigative, nonché lo scambio di dati su persone sospette e sulle organizzazioni criminali operanti nei due territori. I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste, nelle situazioni pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due parti. Alcuni articoli sono quindi dedicati alla protezione dei testimoni e dei loro familiari, ai limiti all'uso dei dati personali e al distacco di esperti per la sicurezza. L'intesa dispone altresì la possibilità per le autorità competenti di concludere accordi di esecuzione, regola la gestione delle spese ordinarie e disciplina le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, la durata, l'entrata in vigore e le modalità per la sua eventuale modifica. II disegno di legge consta di quattro articoli relativi all'autorizzazione, alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del testo. oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 120.000 euro annui. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. L'Accordo, pur in assenza di richiami formali nel preambolo, appare compatibile con gli obblighi internazionali dell'Italia e, in particolare, tiene conto nella sostanza delle disposizioni contenute delle Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo e contro la criminalità organizzata transnazionale. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

nostri lavori, anticipo già in questa sede il voto favorevole della Lega Nord su questo provvedimento, sugli articoli e per il voto finale.

Signor Presidente, non si può non spendere alcune parole per Israele e per gli accordi che stringiamo con questo Paese. Questo Accordo, firmato nel 2013, sostituisce una convenzione precedente del 2005. Esso prevede una spesa complessiva superiore a 120.000 euro. È prevista una serie di corsi di formazione e scambi di informazioni che, a mio avviso, non ha alcuna utilità in Italia, in quanto noi non affrontiamo minacce simili a quelle che affronta Israele né, tantomeno, ci troviamo in presenza di territori morfologicamente omogenei. Risulta poi preoccupante la collaborazione nella gestione dell'ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa. Le nostre forze di polizia sono perfettamente addestrate ad affrontare questo genere di eventi e non si capisce per quale motivo dovremmo spendere altri soldi per cooperare in un settore che riguarda strettamente l'ordine pubblico interno dei rispettivi Paesi. Inoltre, c'è una grande differenza tra i reati che vengono puniti nel Paese mediorientale rispetto a quelli che vengono puniti nel nostro. Per fare solo un esempio, potremmo riferirci alla legislazione penale sui minori, soprattutto palestinesi, rispetto alle tutele previste nel nostro Paese, ma le differenze non si fermano qui, ovviamente. Riteniamo dunque che l'accordo firmato nel 2005 sia già sufficiente a garantire la cooperazione sulla sicurezza dei rispettivi Paesi, senza aggravare lo Stato di ulteriori spese che - ripeto - a nostro avviso sono sostanzialmente inutili in termini sia di aggiornamento del nostro personale, che di minacce che il nostro Paese deve affrontare.

e non c'è dubbio che quando si parla dei temi della sicurezza e della difesa di tutto il mondo, ad iniziare dal nostro Paese, non si può pensare di difendere solo i nostri confini senza immaginare di essere, invece, protagonisti anche dello scenario internazionale. Il voto del Gruppo Area Popolare

gestisce l'emergenza ed il contrasto al terrorismo, agli attentati ed al lancio di missili ogni giorno. È un Paese che ha inventato un sistema di

nonché la gratitudine per l'impegno nella lotta al terrorismo che quel Paese è chiamato a svolgere e che svolge dando a tutti lezione su come lo si deve fare.

Signor Presidente, la Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi. L'intesa ricalca il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, che è stata alla base di molti accordi con altri Paesi, tra cui quello che esamineremo tra poco che riguarda le Filippine, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. L'accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili d'impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili d'impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di un'organizzazione stabile. Quanto agli utili di capitale, la Convenzione stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa. In materia di pensioni, la Convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte. Per i redditi di professori ed insegnanti, l'accordo, per facilitare gli scambi, dispone un'esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgono attività di ricerca o insegnamento. Sono poi previsti il principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione dei conflitti, lo scambio d'informazioni e l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari. Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione e alla ratifica, all'ordine di esecuzione e all'entrata in vigore. Non sono previsti oneri. Il testo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

Signor Presidente, parlando di Barbados vengono in mente il Paradiso: spiagge da sogno, mare cristallino, rigogliosa ed esotica vegetazione. Un posto meraviglioso. Oltre che essere un paradiso per il turismo, è un paradiso fiscale, soprattutto per le imprese di grandi dimensioni. Bisogna innanzitutto distinguere tra le persone fisiche e le società. le società. Le società godono di molti privilegi, come ad esempio: dieci anni di esenzione dal pagamento delle tasse sul reddito, seguiti da una aliquota fissa del 2,5 per cento. Ma fin qui nulla di scorretto, poiché il Paese è molto piccolo e le esigenze di spesa dello Stato sono sicuramente più contenute delle nostre. È proprio il caso di citare un articolo di Valerio Castronovo del 14 agosto 2016 su «Il Sole 24 Ore», dal titolo «È il capitalismo, bellezza», ovvero come giudicare scorretta una concorrenza basata su tasse più basse e servizi alle imprese migliori. Sulla trasparenza bancaria, invece, Barbados è attualmente inserito nelle *black list* degli Stati non collaborativi previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. fa inoltre parte della cosiddetta lista *top* 30 dei paradisi fiscali predisposta dall'Unione europea. Come non concludere che la firma di questo accordo è un passo decisivo verso l'uscita dalla *black list* italiana e ovviamente un'ottima referenza anche per uscire dalla *top list* europea, sempre che ciò sia di interesse per entrambe le parti? È da evidenziare inoltre che rispetto al modello di Convenzione OCSE, comunemente usato dal nostro Paese per siglare accordi di questo tipo, in questo caso ci sono da notare diverse anomalie, come ad esempio: l'articolo 14 stabilisce una corsia privilegiata per le cosiddette stabili organizzazioni, che sarebbero «piattaforma di trivellazione o nave utilizzate per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali» quale stabile organizzazione, «se la durata oltrepassa i sei mesi». La difformità rispetto al modello OCSE riguarda l'articolo 28, che stabilisce la possibilità di rimborsi al contribuente soprattutto nel caso di tassazioni improprie. È inoltre da rilevare che lo Stato caraibico ha recentemente sottoscritto la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza in materia fiscale promossa da OCSE e Consiglio d'Europa, e rientra tra i Paesi che si sono impegnati ad effettuare, entro il settembre 2017, la prima trasmissione di dati secondo il nuovo il nuovo *standard* di scambio automatico OCSE in materia di informazioni finanziarie. Analoghi accordi sono stati sottoscritti anche con gli Stati Uniti. Questo accordo va probabilmente nella giusta direzione, quella di una maggiore trasparenza e di regole certe, tuttavia non è adeguato ad affrontare il prossimo futuro, anche in ragione della trasformazione del mercato finanziario e delle imprese. È un accordo nato già vecchio per molti versi. in ragione della necessità di proseguire un percorso di dialogo e di recuperare base imponibile legittima, seppur in presenza delle perplessità evidenziate, annuncio il nostro voto favorevole.

tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, del 5 dicembre 1980,

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. Il Protocollo in esame è finalizzato ad aggiornare la Convenzione bilaterale risalente al 1980, consentendo di ampliarne il campo di applicazione, includendovi, per l'Italia, anche l'imposta regionale sulle attività produttive. L'articolo III modifica alcune disposizioni della Convenzione vigente, riformulando in particolare quella relativa al metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppia imposizione, rendendola adeguata alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle Convenzioni fiscali. Il medesimo articolo elimina il meccanismo che prevedeva la possibilità per i soggetti italiani che operano nel territorio delle Filippine di attribuirsi il pagamento di imposte virtuali su canoni, interessi o dividendi, anche qualora le stesse non venissero effettivamente prelevate per tali fattispecie reddituali. Il successivo articolo IV amplia la cooperazione fra le amministrazioni, prevedendo fra l'altro il superamento del segreto bancario. L'articolo costituisce dunque la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa fra le Parti in materia di scambio di informazione, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, consentendo al contempo di migliorare la trasparenza dei rapporti fra le autorità fiscali dei due Paesi. Da ultimo, l'articolo V dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo al momento dello scambio delle notifiche delle procedure di recepimento del nuovo accordo nei rispettivi ordinamenti. Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa come dall'introduzione delle disposizioni della Convenzione non dovrebbero determinarsi effetti di gettito per l'erario italiano. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea.

al fine di evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale. Noi condividiamo queste finalità. Oggi abbiamo uno strumento più moderno, più agile e facilmente applicabile che sicuramente porterà a dei risultati migliori; uno strumento maggiormente performante rispetto ai vecchi accordi esistenti. Come dicevo prima, condividiamo le finalità e ci auguriamo che il prima possibile possa trovare applicazione il contenuto di questa ratifica.

sono condivise e soprattutto è uno strumento che può dare risultati migliori rispetto a quello attualmente in vigore.

di martedì 17 gennaio, alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella stessa giornata di martedì.

La Puglia, in special modo, è la Regione in cui le avversità climatiche hanno travolto il territorio che non è riuscito a far fronte all'eccezionalità di questi eventi. Il comparto ortofrutticolo, che rappresenta da sempre un'eccellenza in Italia e nel mondo, è stato messo in ginocchio. Le perdite parziali parlano già di oltre 110 milioni di euro, ma il bilancio è destinato a salire. La Puglia è uno dei principali produttori di ortofrutta a livello nazionale e la diminuzione del quantitativo dei prodotti ortofrutticoli della Puglia provocherà inevitabilmente la scarsità delle materie prime in tutto il Paese, l'aumento dei prezzi dell'approvvigionamento esistente, nonché ricadute occupazionali su tutta la filiera agricola. Il Gruppo CoR ha presentato un'interrogazione per chiedere al ministro Martina di agire con tempestività e presentare un provvedimento che permetta alle aziende agricole di tornare a produrre senza il gravame causato dalle perdite determinate da questi tristi eventi. Auspichiamo, quindi, che il Ministro venga a riferire in quest'Assemblea sulle strategie che il Governo intende adottare per fronteggiare questa situazione. Signor Presidente, colleghi, intervengo in merito alla gravissima situazione in cui si trova il sovrintendente di polizia artificiere rimasto gravemente ferito a Firenze dall'esplosione di un ordigno artigianale la mattina di Capodanno del 2017 (abbiamo iniziato così il nostro anno in Italia). Mario Vece, di 39 anni, ha perso la mano sinistra e quasi totalmente l'occhio destro

probabilmente non l'ultimo, che si è concluso positivamente. Io mi recherò in ospedale per portare la solidarietà mia personale da cittadina di Firenze, ma vi parlo in questa perché da membro del Consiglio di Presidenza vorrei portare anche quella del Senato della Repubblica e sono certa di poter portare anche la vostra, colleghi. Il sovrintendente Mario Vece, infatti, nell'esercizio delle sue funzioni, per garantire la nostra sicurezza è stato vittima di un incidente gravissimo che ovviamente sconvolgerà per sempre la sua vita a quella dei suoi famigliari. Ovviamente sono criminali senza animo i responsabili dell'attentato, persone che ritengono che la lotta politica vada fatta con il sangue e la distruzione, soggetti malavitosi che, secondo le dichiarazioni riportate sulla stampa, come avete visto, farebbero capo ad ambienti anarco-insurrezionalisti che di fatto pensano che la lotta politica vada fatta con il sangue. Le ferite di Mario Vece sono ferite alla democrazia e alle nostre istituzioni. Non sono nuovi questi soggetti; hanno già colpito a Firenze, hanno usato il medesimo sistema di ordigni esplosivi contro sedi sedi dell'organizzazione di estrema destra CasaPound, ma non è questo il punto. Il punto è che la lotta politica deve essere civile. È una lotta che deve essere svolta con le parole, con gli argomenti e non certamente con queste modalità che sono inaccettabili. Concludo qui il mio intervento, Presidente. Volevo sono manifestare la vicinanza del Senato della Repubblica all'artificiere Mario Vece affinché nessuno, nel vortice delle notizie che si sovrappongono giorno dopo giorno, dimentichi la storia di quest'uomo che comunque ha compiuto tale sacrificio per proteggere noi, tutti noi, come tanti poliziotti, come le Forze dell'ordine fanno ogni giorno con un elevato rischio personale. Noi, dopo la notizia, ce ne dimentichiamo, ma in ospedale c'è un uomo che sta soffrendo moltissimo e la sua famiglia, oltretutto, vive a Salerno

di 300.000 abitanti del Veneto. Noi ci battiamo da tre anni perché venga chiuso il rubinetto dell'azienda che inquina, che è stata già da tempo individuata. Però nulla è stato fatto dal Governo, che anzi ha triplicato i valori di soglia, e nulla è stato fatto dal Governo regionale, che anzi ci ha accusato di procurato allarme, minacciando azioni legali nei confronti del Movimento 5 Stelle. Ora, però, sono emersi nuovi dati e nuovi studi gravi e allarmanti. dei nati con peso molto basso, dei nati piccoli per età gestazionali ed alcune malformazioni maggiori tra cui anomalie del sistema nervoso, anomalie del sistema circolatorio e cromosomiche. Nei 21 Comuni interessati nel Veneto si assiste ad un significativo aumento della mortalità. Le patologie associate ai PFAS sono in particolare le cardiopatie ischemiche, per cui la mortalità è aumentata del 21

Addirittura vi è un eccesso significativo di ipertiroidismo. Presidente, in Veneto si sta morendo di PFAS. Non lo diciamo solo noi che bisogna chiudere i rubinetti dell'inquinamento, lo dice Domenico Mantoan, direttore generale della sanità della Regione Veneto che per firmare la sua relazione chiede l'immediata rimozione delle fonti di contaminazione. Per uno scherzo del destino anche lui è vittima di questo inquinamento. Pare che si sia sottoposto o intenda sottoporsi a breve a plasmaferesi: per chi non lo sapesse è il lavaggio del proprio sangue. Peccato che in questa situazione vi siano 300.000 cittadini in Veneto. Veneto. Al governo regionale e nazionale chiediamo per l'ennesima volta di svegliarsi, di rispondere alle interrogazioni che giacciono senza risposta ormai da anni e di intervenire per far chiudere la fonte dell'inquinamento che è stata chiaramente individuata. Chi inquina deve pagare e qui ci sono danni per miliardi e miliardi. Termino, però, con una domanda: chi pagherà per tutte le vite che sono state spezzate perché non si è intervenuti prima per porre fine a questo inquinamento? Presidente, ancora uno scandalo nella gestione dei migranti: il 3 gennaio 2017 le Forze dell'ordine sono intervenute a Cona, in Provincia di Venezia, dopo una rivolta scoppiata in seguito alla morte di una ragazza ivoriana di 25 anni. Il centro è gestito dalla società che - come riporta «Il Fatto quotidiano» - è nome conosciuto per diverse inchieste: truffa, falso e maltrattamenti sono le ipotesi di reato a carico dei vertici della Essa è diventata *leader*, in pochissimi anni, nella gestione del mercato dell'accoglienza, con un fatturato passato da 114.000 euro nel 2011 a quasi 20 milioni di euro nel 2016, dopo esserci aggiudicata importanti strutture in tre Province: Oderzo, Cona Padova. Fino a poco tempo fa, gestiva l'ex caserma Prandina, dove, alle porte del centro storico, sono transitati centinaia di migranti (troppi). Ho visitato quella tendopoli e ho presentato un atto di sindacato ispettivo che ancora non ha avuto risposta. Il caso è così lampante, signor Presidente, che Ugo Campagnaro, presidente regionale di Confcooperative, ebbe a dichiarare che questo è un sistema che non risponde alle logiche della buona accoglienza, della qualità dell'intervento, dell'integrazione e della relazione. Si tratta invece di un modello che guarda soprattutto al *business*, prendendo le distanze da quel soggetto gestore e dalla maniera in cui operava. Negli anni Ecofficina è stata oggetto di inchieste giornalistiche che riportano gli intrecci parentali con la politica. è Gaetano Battocchio, mentre l'amministratore delegato è Sara Felpati, moglie di Simone Borile, ex presidente del Consorzio Padova Sud e vicepresidente della controllata Padova Tre, le stesse in cui lavorano o hanno lavorato, tra gli altri, Francesca Degani, sorella di Barbara, ex presidente della Provincia e Sottosegretario all'ambiente con il Nuovo Centrodestra, ma anche Emiliano Manzato, figlio di Sergio, ex deputato dei DS e sindaco di Stanghella. E poi una pletora di parenti di politici locali: mogli, figli e cognate di assessori, vicesindaci, consiglieri comunali di destra, sinistra e centro. L'unione tra Padova Tre ed Ecofficina, oggetto di indagini giornalistiche, si sarebbe conclusa nel 2014, ma i loro legami sono finiti ancora al centro di un'inchiesta del pubblico ministero di Padova Federica Baccaglini su un buco in bilancio da 30 milioni di euro. nel novembre scorso gli uomini della Guardia di finanza sono arrivati a perquisire gli uffici di Ecofficina per un sospetto scambio di denaro tra le casse della Coop e quelle della società di raccolta rifiuti. presentato un ulteriore atto di sindacato ispettivo, in cui chiedo di sapere quali informazioni il Governo abbia in riferimento alla morte della ragazza presso il centro di accoglienza e sulla rivolta scoppiata; quali iniziative abbia in animo di adottare per verificare ed eventualmente risolvere le criticità evidenziate; come voglia prevenire la gestione di questi centri di accoglienza da parte di soggetti che non abbiano gli *standard* doverosi di qualità e dignità negli interventi; se intenda attivare un sistema di monitoraggio adeguato; infine

Presidente, ieri abbiamo avuto modo di conoscere dalle cronache giornalistiche un nuovo episodio della gestione della ricostruzione post terremoto secondo

Credo che questo sia il fallimento totale di qualsiasi scelta politica seria di risposta a questa emergenza, che - lo ricordo - nei mesi passati ha visto sfilare

che ci sia stato un sorteggio. Dopo la disgrazia, dopo la malasorte, adesso ci si deve affidare alla buona sorte. Ma questa non è una modalità seria con cui operare. Non è possibile che si proceda con questa modalità nei confronti di gente che ancora oggi aspetta sotto le tende e sotto la neve. La cosa ancora più raccapricciante è che ci si affidi alle raccolte di fondi privati, quando ci sono centinaia di milioni che dovrebbero essere a disposizione e quando purtroppo - lo dico per l'ennesima volta - la burocrazia sta vincendo sul buonsenso.

Sono veramente rammaricato e non dico altro perché vorrebbe dire scadere nel contenuto. Nei prossimi giorni tornerò ancora in quelle case e tra quella gente

avverrà, avremo abdicato al nostro ruolo. Questo non possiamo permettercelo; noi non lo permetteremo.

il parco archeologico di Liternum, nel Comune di Giuliano, in provincia di Napoli.

dell'aria. Abbiamo avuto la brillante idea di riaprire una centrale a carbone. Sappiamo tutti che il carbone è il combustibile del futuro: sicuro, pulito ed economico (naturalmente sono sarcastico). Abbiamo riaperto una centrale a Genova perché la Francia produce meno energia con il nucleare. Noi italiani siamo stati bravissimi negli anni passati: abbiamo aumentato notevolmente la nostra produzione da rinnovabili e, quindi, siamo tranquilli (anche qui sono tristemente sarcastico). L'Italia negli ultimi due anni è in retromarcia. Colleghi della maggioranza, per favore mettetevelo in testa. Sono dati ufficiali: due anni fa abbiamo perso il 5 per cento di elettricità da rinnovabili e l'anno scorso il 2 per cento. Siamo in retromarcia,

non ha più alcuna remora. Ha rilasciato un'intervista a «Popular Science», che vi invito a leggere, nella quale sposa completamente rinnovabili ed efficienza. Come potrebbe essere altrimenti

Vorrei invitare tutti ad andare in miniera a estrarlo per capire cosa comporta. È un messaggio per tutti gli italiani.